Onorevoli co1leghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente. Nella giornata di oggi si discuterà il disegno di Legge comunitaria 2008. Domani mattina saranno poste all'ordine del giorno mozioni sugli ammortizzatori sociali. I Gruppi potranno intervenire per 20 minuti ciascuno, comprensivi di interventi in discussione generale e dichiarazione di voto. Gli illustratori delle mozioni presentate avranno a disposizione 5 minuti ciascuno. A conclusione di tale dibattito saranno discusse le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri. È stato poi approvato il calendario delle prossime due settimane, fino a giovedì 26 marzo. Nella seduta pomeridiana di martedì 17 e in quella antimeridiana di mercoledì 18, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi nel corso di questa settimana (Legge comunitaria 2008 e ratifiche di accordi internazionali), sarà discussa la mozione Tomassini - ed altre analoghe eventualmente presentate - sulla lotta contro l'AIDS. Si svolgerà inoltre un dibattito sugli strumenti della legislazione, che si concluderà senza votazione di strumenti di indirizzo. Per entrambi i dibattiti i Gruppi avranno a disposizione 20 minuti ciascuno. In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 18 marzo la Presidenza ricorderà la figura di Chiara Lubich ad un anno dalla sua scomparsa. Successivamente potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi. nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo inizierà l'esame dei disegni di legge sul testamento biologico, nel testo definito dalla Commissione o comunque nel testo base del relatore. In tale seduta saranno discusse eventuali questioni incidentali e si passerà poi alla discussione generale che si concluderà entro la giornata di giovedì 19. Per tale fase, al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, non si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul testamento biologico, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, ove la Commissione concluda i propri lavori entro la giornata di domani, giovedì 12 marzo, gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 13; qualora la Commissione concluda invece nella giornata di venerdì, il termine è fissato per le ore 15 di lunedì 16 marzo. Le votazioni sugli articoli e sugli emendamenti avranno inizio nella seduta antimeridiana di martedì 24 marzo e proseguiranno nelle sedute successive fino al pomeriggio di giovedì 26. Per la fase delle votazioni, i tempi sono stati ripartiti per complessive 18 ore, escluse le dichiarazioni di voto finali. Il calendario potrà essere integrato con l'esame di decreti-legge già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati. Come già annunciato, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana successiva alle festività pasquali (dal 14 al 17 aprile). Le Commissioni potranno peraltro convocarsi in relazione ai rispettivi programmi di lavoro.

Voglio fare anche una premessa. Poiché con molta cortesia il ministro Vito mi aveva dato un'interpretazione - mi pare sposata anche dal presidente Gasparri - circa l'autenticità delle dichiarazioni riportate dalle agenzie, e quindi l'autenticità dell'interpretazione da dare alle parole del Presidente del Consiglio, ho avuto cura di riscontrare il video, anche perché talvolta, come si suol dire, si sente ma non si crede che ciò che si sta sentendo possa essere vero. Non ho alcun dubbio, dunque, a questo punto, né sull'autenticità delle parole attribuite al Presidente del Consiglio, e riportate dalle agenzie di stampa, di stampa, né sulla genuinità della loro interpretazione. Peraltro, colleghi, le abbiamo lette tutti. Ciò che il Presidente del Consiglio propone non è un'innovazione regolamentare che valga a rendere più efficiente il lavoro del Parlamento, celebrandone quindi la centralità, peraltro in una democrazia parlamentare come la nostra; se così fosse, avremmo potuto molto più ragionevolmente affidarci alle proposte di modifica dei Regolamenti parlamentari presentate da maggioranza e opposizione in discussione alla Giunta per il Regolamento. No, il problema del Presidente del Consiglio è che dopo 70-80 votazioni una persona che non è tuttologa possa anche deprimersi; meglio ancora, i nostri deputati sono persone del fare e non funzionari di partito che si deprimono in Parlamento con votazioni continuative. Ciò che si rivela in tutta chiarezza, Presidente, non è un dibattito di natura costituzionalistica e con ricaduta regolamentare sui meccanismi che meglio regolano l'attività legislativa e la rendono più efficiente, ma il fatto che il Presidente del Consiglio, che porta in Parlamento persone del fare che si scocciano a stare in Parlamento a discutere provvedimenti e ad esprimere il proprio voto ricordandosi che ogni parlamentare rappresenta la Nazione, propone propone - ovviamente - non una riconduzione a ragione dei Regolamenti parlamentari o dell'esercizio della funzione parlamentare, ma del Parlamento medesimo. Signor Presidente, la cosa non ci stupisce perché il presidente Berlusconi ancora una volta dimostra il grande disprezzo (ovviamente lo fa con l'eleganza che gli è consueta), la sufficienza con cui guarda al cuore della democrazia italiana.

inconsapevole della gravità delle sue affermazioni (perché per esserne consapevole avrebbe dovuto avere alle spalle una cultura istituzionale che non possiede e che comunque sarebbe un requisito esigibile da parte di chiunque nei confronti di chi esercita le funzioni di Presidente del Consiglio, e se non ci crede deve almeno fare finta di crederci, secondo me), in Senato una discussione sulla decretazione d'urgenza, altro aspetto di quella disistima nei confronti del Parlamento o meglio di quella incomprensione delle ragioni profonde per le quali una democrazia come la nostra sul Parlamento si fonda. Mi chiedo, in questo quadro, che cosa c'entri la discussione sui Regolamenti parlamentari, che invece c'entrava eccome e ben a ragione, perché è interesse di tutti, maggioranza ed opposizione, fare in modo che i Regolamenti parlamentari assecondino una capacità del Parlamento di rispondere con tempestività ed approfondimento alla richiesta di decisione politica che sale dal Paese. Mapotremmo aggiungere altro, perché nelle dichiarazioni di ieri il presidente Berlusconi ha fatto ancheriferimento a una proposta di iniziativa popolare con la quale si riduca a metà il numero dei parlamentari.

di non prenderci in giro, perché se il Presidente della più grande forza politica del Paese, capo della maggioranza, Presidente del Consiglio, si inventa una legge di iniziativa popolare pur avendo tutti gli strumenti per portare immediatamente in Parlamento tale questione, con l'autorità della sua maggioranza e del suo Governo, questo serve forse a buttare fumo negli occhi degli allocchi, ma non credo che possa essere considerata da parte dei parlamentari - e dei parlamentari dell'opposizione - una proposta che abbia un minimo di fondamento. Anche questo, signor è il segnale di un modo demagogico, populistico, strumentale e sprezzante nei confronti delle forme democratiche con cui ordinariamente il Presidente del Consiglio si rivolge al Parlamento e agli italiani e alle italiane.

Ma noi abbiamo il dovere, maggioranza e opposizione, di mantenere vigile - ripeto, vigile - la consapevolezza negli italiani e nelle italiane che in questo luogo, almeno in questo luogo, qui al Senato c'è la possibilità di rappresentare gli interessi di tutti coloro i quali attraverseranno con difficoltà e con sacrificio la crisi, senza che ciò costi un grammo di democrazia al nostro Paese, se vogliamo ritrovare il nostro Paese intatto e capace di rimettersi in piedi quando tutto questo finirà.

una visione disincantata e preoccupata delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Disincantata perché ovviamente la sua opinione sul ruolo delle istituzioni e della politica è nota da più di un decennio

Noi siamo d'accordo con la collega Finocchiaro affinché venga immediatamente calendarizzata la proposta di legge costituzionale per la riduzione del loro numero. Considerato che siamo tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, non si vede la ragione per la quale, anziché affrontare in con concretezza e serietà il tema della riduzione del numero dei parlamentari (avendo peraltro una maggioranza così larga che consente una modifica costituzionale rapida), si debba fare ricorso ai gazebo della libertà per discutere di questo tema. In realtà è il Parlamento che deve votare una legge costituzionale. Facciamolo, ma con serietà, evitando di dire altro.

Manca all'appello solo l'aspetto del voto delegato. Ebbene, non voglio fare il sindacalista dei Capigruppo, ma personalmente non credo sia opportuno né costituzionalmente orientato un giudizio in forza del quale si immagini che i Capigruppo possano assumersi la responsabilità per ciascun parlamentare, considerato il principio costituzionale del divieto di mandato imperativo. Ma non è questo, signor Presidente. Credo che tutti questi argomenti, proprio per il disincanto che abbiamo rispetto al modo in cui vengono esternati dal Presidente del Consiglio, debbano essere ricondotti nelle sedi proprie, a cominciare dal dibattito che la prossima settimana avremo sulla posizione del Presidente del Consiglio e del Governo in merito all'uso della decretazione d'urgenza. È quella la sede in cui anche il Presidente del Consiglio dovrà riferirci

Ma noi siamo preoccupati, signor Presidente, per una ragione molto semplice: agitare questi argomenti, peraltro fuori dalle sedi proprie (quindi con la consapevolezza che non verranno mai affrontati, ma è bene dirlo perché si

economica non intendiamo fare sconti. Pertanto affronteremo in un dibattito la visione del Governo e del Presidente del Consiglio sulla democrazia e su come sta funzionando il Parlamento, ma vogliamo che il Paese e i cittadini siano concentrati sulla capacità che questo Governo ha o non ha di produrre provvedimenti buoni per le famiglie e le imprese italiane. Questo ci interessa in questa fase. Siamo più interessati a che il Governo ci riferisca in merito e anche in tempi rapidi, come accadrà domani con le mozioni che abbiamo presentato. Presidente, colleghi, non vogliamo dire di avere il *copyright* su tutto ciò che abbiamo ascoltato: conosciamo da tempo, e le abbiamo ricordate anche in questa Aula, le pulsioni non propriamente parlamentariste del presidente Berlusconi, che per sua scelta si distingue per una cronica assenza dalle sedute del Senato e anche della Camera. Vedete, quanto è successo ieri non è il frutto della fantasia delle opposizioni: il Presidente del Consiglio,

Voglio ricordare, in merito, un precedente democratico, quello dell'Assemblea nazionale del popolo della Cina popolare, che nel 1982,

L'Italia è un Paese diverso. È un Paese nato dalla Resistenza, con una democrazia consolidata, che non può essere insultata da dichiarazioni estemporanee del Presidente del Consiglio. *Stop and go*, afferma e poi ritira, afferma e poi ci sono gli interpreti autentici del suo ragionamento. Non va bene, signor Presidente del Consiglio: ce lo venga a dire in quest'Aula che non dobbiamo più votare. Ce lo venga a dire in quest'Aula che non è ammesso neppure il voto elettronico

sfidare il Presidente del Consiglio in Aula ad un dibattito serio su questi temi, non con le chiacchiere. Sono pendenti disegni di legge costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari. La legge di iniziativa popolare è un volgare mezzuccio per ingannare mediaticamente il Paese, ma, inganna oggi inganna domani, il Paese capisce e capirà ancora meglio nei prossimi mesi.

in via trasversale il valore e l'orgoglio del Parlamento repubblicano. Poi valuteremo gli strumenti perché il Parlamento sia più snello nelle decisioni e più pronto nell'approvazione delle leggi. Dobbiamo però far salva la democrazia nel nostro Paese, che, a furia

Signor Presidente, francamente ho trovato esagerati, anche nei toni, gli interventi della senatrice Finocchiaro e del collega Belisario. Ognuno svolge il suo ruolo. Ieri il presidente Berlusconi, anche attraverso una provocazione, ha voluto ribadire la necessità per il Governo di riuscire ad intervenire nell'attività legislativa del Parlamento con tempi certi. Questa è una necessità che di fatto, più volte, anche i Gruppi dell'opposizione hanno manifestato di condividere.

richiesto un *referendum* che non ne ha permesso l'approvazione. Noi il numero dei parlamentari - non a parole, non presentando proposte di legge che poi non sono state votate - lo abbiamo davvero ridotto in Parlamento Parlamento e vogliamo farlo anche in questa legislatura. Le riforme istituzionali calendarizzate in 1a Commissione, che andranno a ridurre il numero dei parlamentari, a finirla per sempre con questo bicameralismo perfetto che ingolfa la produzione legislativa in Parlamento e a creare finalmente un Senato federale, sono una priorità di questo Governo e di questa maggioranza. Dunque, al di là delle parole bisogna vedere i fatti, e noi li abbiamo realizzati. Siamo stati gli unici a ridurre il numero dei parlamentari in Parlamento, ma voi ce lo avete impedito attraverso il *referendum* e la campagna contro la legge che avevamo approvato in Parlamento, impedendo di fatto la riduzione del numero dei parlamentari.

Signor Presidente, colleghi, non mi meraviglia l'enfasi dei toni che sono stati usati dalla presidente Finocchiaro su un tema certamente delicato, ma ho apprezzato di più le considerazioni che ha svolto poc'anzi in quest'Aula il presidente D'Alia.

(ve n'è traccia anche nelle dichiarazioni e nelle interviste riportate dai giornali di oggi), perché è evidente che un'innovazione come quella di affidare il voto solo ai Capigruppo richiederebbe particolari procedure e condivisioni,

un'ampia, organica, seria riforma della Costituzione che affrontava e risolveva i temi del federalismo, del bicameralismo e della riduzione del numero dei membri del Parlamento: una decisione coraggiosa, non teorica e propagandistica, ma approvata con una doppia lettura

torneremo a discuterne, nel rispetto delle istituzioni parlamentari e anche alla luce di una visione più equilibrata. La riforma del federalismo e la necessità di meccanismi di decisione più snelli portano con sé anche il problema della riduzione del numero dei parlamentari, su cui già ci siamo cimentati ed espressi, e voi siete stati sempre dall'altra parte. Questa è la verità dei fatti, dei numeri, dei voti del Parlamento, dell'espressione di volontà nei *referendum*.

alla Presidenza del Senato. Ne abbiamo parlato poco fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo: vogliamo sapere quale sarà lo sviluppo del dibattito sulla riforma del Regolamento.

L'alternativa alla decretazione d'urgenza, l'alternativa ad alcuni strumenti il cui uso, a volte, può apparire eccessivo è la possibilità di decidere, perché il più grande vincolo di una democrazia è la volontà popolare degli elettori,

tutti i parlamentari e tutte le realtà del territorio, devono però portare a decisioni e a votazioni, non a lungaggini, all'ostruzionismo o a riti che a volte impediscono ai cittadini di vedere risolti i problemi del lavoro, della sicurezza, della famiglia, della casa. Credo che le maggioranze che di volta in volta il corpo elettorale indica con la sua libera espressione di voto debbano avere il diritto di governare un Paese. La vera risposta ad una sana provocazione che ci fa discutere di questi argomenti, dunque, è una moderna riforma dei Regolamenti, è la realizzazione di un'autentica democrazia decidente. Per quanto riguarda la riduzione dei membri del Parlamento e altre questioni, presidente Finocchiaro, vi aspettiamo alla prova dei fatti, quando ne discuteremo e conteranno i voti espressi da tutti i parlamentari in Aula.

Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge comunitaria per il 2008 è stato presentato il 6 ottobre scorso, scontando purtroppo il periodo di inattività dovuto allo scioglimento anticipato delle Camere. Il precedente Governo, infatti, aveva già presentato all'inizio dell'anno, come previsto dalla legge n. 11 del 2005, un disegno di legge comunitaria, che non ha potuto essere esaminato proprio a causa dell'interruzione della legislatura. Successivamente, per motivi di urgenza, ad aprile è stato emanato il cosiddetto decreto salva-infrazioni (decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59), ma il nuovo disegno di legge comunitaria, che in buona parte riproduce i contenuti di quello precedente, è stato presentato al Parlamento nel mese di ottobre. Oggi esso giunge all'attenzione dell'Assemblea del Senato dopo cinque mesi di esame in Commissione, con più di 180 tra emendamenti e subemendamenti - molti di iniziativa dello stesso Governo - attraverso i quali il testo del provvedimento ha visto quasi raddoppiare il numero dei suoi articoli. Questi dati danno anzitutto la misura della mole delle disposizioni comunitarie che occorre recepire e, in qualche modo, anche delle difficoltà che il nostro ordinamento incontra nel dare piena e corretta attuazione al diritto europeo. L'Italia continua infatti a figurare tra i Paesi con il maggior numero di procedure di infrazione a suo carico, anche se la tendenza di questo ultimo periodo è sicuramente molto positiva: dagli ultimi dati resi disponibili dal Dipartimento per le politiche comunitarie, aggiornati al 19 febbraio scorso, risultano aperte 164 procedure di infrazione (contro le 237 del 2007), di cui 136 per non corretta attuazione e 28 per mancata trasposizione. Lo strumento della legge comunitaria annuale, introdotto con la legge La Pergola, poi abrogata e è da molti, in Italia e in Europa, considerato come un ottimo modello giuridico per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Ribadita la bontà di questo strumento, esso presenta tuttavia alcuni inconvenienti, soprattutto dal punto di vista delle procedure parlamentari vigenti, a cui sarebbe opportuno ovviare. Uno dei punti principali è contenuto nell'articolo 144-*bis*, nella parte in cui dispone che il disegno di legge comunitaria sia discusso congiuntamente alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Sulla base di questa norma, l'Aula del Senato si trova oggi a esaminare la relazione annuale relativa al 2007 - di cui è relatrice la senatrice Licastro Scardino - dopo più di un anno dalla fine di quello a cui si riferisce, per non parlare dell'altro ramo del Parlamento che deve aspettare la fase della seconda lettura. Tale problematica temporale, unitamente alla considerazione della diversa natura tra i due atti (la relazione più di carattere politico‑programmatico e più attinente alla fase ascendente, la legge comunitaria relativa esclusivamente alla fase discendente), hanno suggerito già da diversi anni l'opportunità di svincolare l'esame della relazione annuale da quello del disegno di legge comunitaria ed eventualmente abbinarlo all'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Consiglio. Le relazioni annuali (intendo tutte), a causa dei motivi sopraesposti, mancano di incisività e vengono meno a quell'aspetto di programmazione politica che sarebbe invece indispensabile per incidere sulla fase ascendente dei provvedimenti «europei», cioè nella fase della formazione delle direttive che, a mio parere, deve diventare la fase cui guardare con maggiore attenzione, perché è in quella fase che bisogna intervenire per incidere veramente sul diritto comunitario. In attesa della definiva approvazione del Trattato di Lisbona, stiamo già sperimentando la possibilità di esaminare le proposte di direttive e trasmettere alla Commissione i pareri, espressi separatamente, dei due rami del nostro Parlamento.

La finalità è quella di fare in modo che il disegno di legge comunitaria annuale, che per legge deve essere presentato entro il mese di gennaio, possa giungere alla sua definitiva approvazione al massimo entro l'autunno dello stesso anno, anche per consentire poi l'esame dei documenti di bilancio. Il disegno di legge comunitaria in esame è passato dai 26 articoli iniziali agli attuali 49 articoli. Per brevità, non mi soffermerò a illustrare tutte le disposizioni, articolo per articolo, limitandomi a evidenziare solo alcune delle importanti normative comunitarie di cui si prevede il recepimento. L'articolo 41, introdotto in Commissione su sollecitazione anche dei senatori di opposizione, reca una delega al Governo per dare attuazione alla direttiva servizi, che avrà un impatto notevole - a mio avviso straordinario - sull'ordinamento, in quanto dovrà assicurare la necessaria omogeneità della regolamentazione dei servizi esclusi quelli di interesse generale come definiti dallo Stato - rispetto ai criteri imposti dalla direttiva, al fine di consentire la mobilità transfrontaliera delle prestazioni e dei prestatori di servizi. La direttiva prevede l'adozione di una serie di misure concrete come la creazione di sportelli unici nazionali per i prestatori di servizi, l'utilizzo sempre più capillare delle procedure elettroniche e la cooperazione amministrativa tra enti, anche di diversa natura, al fine di arrivare ad una semplificazione delle procedure e delle formalità. Tra le modifiche approvate dalla Commissione rispetto ai criteri di delega proposti dal Governo figura anche l'aggiunta della lettera *q)*, finalizzata a garantire l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri. Il Capo III (articoli da 43 a 45) è interamente dedicato ai cosiddetti GECT (gruppi europei di cooperazione territoriale transfrontaliera): le norme previste, necessarie a dare concreta attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006,

Gli articoli da 46 a 49 dettano disposizioni per dare attuazione alle decisioni quadro in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, di scambio di informazioni e di *intelligence* tra le autorità degli Stati membri e di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Quest'ultima direttiva, in particolare, è stata introdotta con un emendamento presentato dal Ministro per le politiche europee il 25 febbraio scorso e consente allo Stato membro che emette una sentenza di condanna definitiva nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro di far scontare la pena nello Stato membro di cittadinanza o di espulsione. Oltre al recepimento di direttive, regolamenti o decisioni quadro che - ripeto - non sto ad elencare, rimandando alla relazione fatta in Commissione e alla lettura del testo, nel disegno di legge sono state introdotte anche molte norme necessarie a dare esecuzione a sentenze della Corte di giustizia o a risolvere procedure di infrazione. Fra queste segnalo l'articolo 18 in materia di caccia, nonché l'articolo 24 in materia tributaria e di giochi *on line*. In conclusione, considerata la natura periodica dello strumento della Legge comunitaria annuale e le importanti ed urgenti disposizioni che esso contiene, mi auguro che il disegno di legge in esame possa giungere alla sua definitiva approvazione il prima possibile,

giunge all'esame dell'Assemblea solo nel 2009, dopo quasi un anno e mezzo dalla fine dell'anno a cui si riferisce e ampiamente dopo la fine dell'anno a cui è riferita la sua parte programmatica, vanificando così ogni sua utilità come strumento di controllo e indirizzo. Pur tenendo conto del periodo di interruzione dei lavori parlamentari, dovuto alla fine della legislatura e alle elezioni per quella corrente, è del tutto evidente la necessità di rivedere il sistema procedurale previsto dal Regolamento del Senato per la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento, in modo svincolato rispetto al disegno di legge comunitaria ed eventualmente concomitante con l'esame dei documenti annuali programmatici dell'Unione europea. Su questo tema la 14a Commissione ha presentato una proposta di modifica alla Giunta per il Regolamento che va nel senso della disgiunzione dell'esame della Relazione annuale e del disegno di legge comunitaria. Nonostante il predetto sfasamento temporale, l'esame della Relazione annuale, nella 14a Commissione, è stato comunque approfondito e utile, anche al fine di dare al Governo opportune indicazioni per migliorarne e valorizzarne le le caratteristiche di uno strumento di bilancio consuntivo e programmatico della politica europea dell'Italia. In particolare, è stata sollevata la necessità di assicurare un maggior raccordo con le relazioni degli anni precedenti, sia nel dare conto delle politiche comunitarie e dell'azione svolta dal Governo, sia nelle rispettive indicazioni programmatiche. In questo senso è stata espressa anche l'esigenza di una maggiore esplicitazione della posizione e dell'opinione del Governo sui singoli argomenti di maggiore interesse per il nostro Paese. L'esame approfondito, svolto anche dalle altre Commissioni in sede consultiva, è stato fonte di numerose indicazioni, che sono state formulate nei rispettivi pareri indirizzati alla 14a Commissione. Per quanto riguarda l'illustrazione del contenuto del documento, rinvio alla relazione contenuta nello stampato all'esame di quest'Aula, limitandomi ad evidenziare che la Relazione annuale è suddivisa in sei parti: la prima tratta del processo d'integrazione e di allargamento; la seconda si concentra sulle prospettive economiche e sulle misure adottate dal Governo nell'ambito della Strategia di Lisbona; la terza è incentrata sulle attività di Governo connesse alle fasi ascendenti e discendenti della normativa comunitaria; la parte quarta quarta tratta del mercato interno e della concorrenza, con particolare riferimento alle quattro libertà di circolazione (dei beni, dei servizi, dei lavoratori e dei capitali), alle liberalizzazione, agli aiuti di Stato, alla tutela della proprietà intellettuale e alla protezione dei consumatori; la parte quinta si sofferma sulle politiche comuni in tema di agricoltura, trasporti, telecomunicazioni, energia, ambiente, fiscalità, coesione, fondi strutturali e lotta contro la frode; infine, la parte sesta si sofferma sulle politiche sociali, offrendo un quadro completo delle iniziative in fase ascendente e discendente, per quanto concerne, tra l'altro, le politiche per la famiglia, per lo sport, per il lavoro, per la salute e per l'istruzione e la formazione. *(Applausi Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, con questo disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione dell'adeguamento del nostro ordinamento al diritto comunitario.

e donne in materia di occupazione e d'impiego entro il 15 luglio 2009 con l'emanazione di un apposito decreto legislativo che permetta l'attuazione della direttiva 2006/54/CE (rifusione di più direttive e trattati, entrati già in vigore a partire dal 1976). un fattore che non ci possiamo più permettere che continui ad essere trascurato, anche in considerazione del fatto che, già con la ratifica del Trattato di Lisbona, ci siamo assunti il compito di prevedere politiche europee, coordinate con esperti di economia e di *welfare*, che pongano le donne al centro di un percorso di innovazione e di crescita. Spesso si dimentica che in Europa hanno diritto al voto 26 milioni di donne e 24 milioni di uomini, così come il fatto che molte delle imprese guidate da donne risultano le più capaci a resistere in fasi - come quella attuale - di profonda crisi economica. A metterlo in evidenza è stata di recente proprio una rilevazione effettuata da Unioncamere e da Infocamere, in base ai dati presenti nel registro delle imprese delle Camere di commercio; paradossalmente, però, alla fine risulta la donna lavoratrice il soggetto complessivamente più danneggiato. Se la donna lavora, entra più ricchezza in famiglia, a patto che ci sia un sistema di servizi sociali adeguato, aumenta il reddito e vi è anche un incremento delle nascite: questo era il punto cardine intorno al quale, a marzo del 2000, a Lisbona i Paesi europei decisero un Piano sull'occupazione femminile, intesa appunto non solo come una questione di genere, ma come volano per l'economia nazionale, che prevedeva di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo del 60 per cento di donne occupate con un lavoro autonomo o dipendente, avendo ben capito che più donne in economia sono la vera innovazione per lo sviluppo del mercato. La media europea di occupazione attualmente si aggira intorno al 54,4 per cento, mentre quella italiana sul 46,3:

La Danimarca guida la classifica con una percentuale quasi irraggiungibile del 73,4 per cento di donne occupate. Il nostro Sud è il luogo europeo dove le donne risultano meno occupate. Le percentuali sono bloccate al 34,7 Dal 1993 al 2006 le occupate sono cresciute di 1.469.000 unità nel centro-nord e solo di 215.000 nel Sud. Molte giovanissime addirittura smettono di cercare lavoro. Le chiamano le "inattive" e sono più di 110.000. Tra i 35 e i 44 anni 8la fascia di maggiore occupazione) al Nord lavorano 75 donne su 100, al centro 68 su 100, al Sud 42 su 100. anche quando arrivano in posizione apicale è comunque destinato loro uno stipendio inferiore di un quarto rispetto a quello del collega uomo. I dati della Presidenza del Consiglio ci dicono che una dirigente guadagna il 26,3 per cento in meno di un collega uomo e questo differenziale retributivo di genere è pari al 23,3 per cento, per cui una donna percepisce, in eguale posizione professionale, tre quarti di uno stipendio in meno rispetto al suo collega, e questo solo nel pubblico. Nel privato la situazione è addirittura peggiore. I dati mostrano che il differenziale di reddito tra uomini e donne è maggiore nelle professioni più qualificate e meglio retribuite, e nelle aree geograficamente dove il reddito medio è più elevato, che risultano essere ancora quelle in fascia di attività femminile già al livello degli obiettivi Lisbona 2010. Non sembra che attualmente il mercato del lavoro, sia nel pubblico che nel privato, offra alle donne un ambiente che garantisca criteri meritocratici né un'adeguata motivazione. per cento delle aziende quotate, escluse banche e assicurazioni, non c'è una donna nei consigli di amministrazione. Su 2.217 consiglieri sono 110 le donne, per cento. Va ancora peggio nelle banche, dove su un campione di 133 istituti di credito, il 72,2 per cento dei consigli di amministrazione non conta nemmeno la presenza di una donna. Benché il 40 per cento dei dipendenti delle banche siano donne solo lo 0,36 per cento ha la qualifica di dirigente, contro il 3,11 degli uomini. C'è qualcosa che non torna visto che a scuola, nelle università, nei concorsi, le votazioni migliori sono sempre quelle delle studentesse.

In politica, poi, la situazione è nota: donne Ministri e Sottosegretari sono soltanto il 20 per cento, le deputate solo il 17 per cento. In questo quadro è dunque necessario ripensare le strategie di sviluppo occupazionale e di partecipazione sociale del soggetto femminile, la cui presenza nel mondo del lavoro è quanto mai strategica per l'implementazione di capitale sociale dei territori, attraverso quindi interventi non solo finalizzati a sostenere un soggetto svantaggiato, ma a valorizzare la donna, che oggi appare come un attore privilegiato perché portatrice di valori essenziali per un effettivo processo di cambiamento economico e sociale. Affinché questo diventi possibile, occorre sostenere un insieme di interventi che tengano conto delle interazioni tra mondo del lavoro, sfera privata, territorio e che permettano di sviluppare politiche e pratiche di flessibilità, costruite su un sistema di tutele sociali e di coesione sociale, che comprendano interventi nel mercato del lavoro, della sicurezza, della vita sociale e familiare, nelle modalità organizzative gestionali delle singole aziende, così come dei servizi territoriali e di conciliazione familiare. Tener conto di tutti questi fattori vuol dire essere in grado di attuare un vero sistema di conciliazione in termini di parità di genere tra la vita lavorativa e quella familiare e quindi su tutte quelle che devono essere le nuove politiche del *welfare* della nostra Nazione e dei nostri territori.

Dato il tempo limitato, mi soffermerò su una questione collegata, oggetto di tante discussioni in questi giorni, e cioè sul fatto che l'Europa preme sull'Italia perché sia uniformata l'età pensionabile in quanto, sul piano dei diritti, considera considera discriminante che le donne vadano in pensione a 60 anni e gli uomini a 65. In teoria, la soluzione potrebbe essere anche quella di abbassare l'età pensionabile degli uomini, ma la situazione dei conti pubblici, in realtà, non ce lo consente e la scelta è quella di elevare l'età delle donne, anche per permettere - così spiega l'Unione europea - un ampliamento delle risorse a favore degli ammortizzatori sociali per i disoccupati. Il Ministro della funzione pubblica ha affermato che «è necessario porre al centro dell'agenda politica l'obiettivo della perequazione verso l'alto dell'età pensionabile di maschi e femmine», che «occorre uscire dall'ipocrisia» e che «se affermiamo che l'invecchiamento attivo è un obiettivo di bene pubblico, è necessario che tutti insieme ci applichiamo per raggiungere questo obiettivo». Peccato che il Governo si sia dimenticato di dire che l'Europa da tempo chiede all'Italia di portare al 60 il livello di occupazione femminile entro il 2010, livello che attualmente è fermo al 43 per cento (e al Sud è anche inferiore), collocando il nostro Paese tra gli ultimi della Comunità, fatto che genera un rilevante spreco di creatività ed abilità. Sappiamo tutti molto bene che in Europa esiste una questione di sostenibilità per i sistemi pensionistici, pensionistici, che tuttavia non può essere risolta con un approccio solo ragionieristico: ed un atteggiamento solo ragionieristico non può e non deve valere né per le donne, né per gli uomini. Comunque, alla fine, chi paga di più sono ancora una che subiscono, da sempre, una situazione di forte svantaggio. Sappiamo inoltre che per le donne è molto difficile competere nel mondo del lavoro, non solo per un retaggio storico ancora non del tutto superato, ma anche perché sulle donne continua a gravare gran parte del «peso» della conduzione familiare, peso che aumenta sensibilmente al momento che si presenta una qualsiasi difficoltà (handicap, anziani non autosufficienti, problemi economici e così via). Sappiamo che il lavoro delle donne è ancora sottopagato, mediamente di circa il 20 per cento, rispetto a quello di un uomo. Se vogliamo davvero favorire la parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego occorre mettere in campo azioni concrete volte al raggiungimento degli obiettivi previsti per l'accesso al lavoro dalla Strategia di Lisbona per il 2010. Anche questa è una rilevantissima indicazione europea. Occorre mettere in campo azioni volte a garantire le carriere delle lavoratrici; occorre contrastare l'espulsione femminile dal mondo del lavoro quando i tempi si fanno difficili essere azioni volte a garantire pari dignità al momento del possibile reimpiego; occorre creare adeguati servizi di sostegno alla maternità ed alla famiglia, senza i quali, di fatto, la donna continua ad essere svantaggiata nelle sue possibilità di accesso al lavoro; occorre tutelare e promuovere le pari opportunità sul piano civile, ma anche e soprattutto su quello culturale, favorendo la formazione, l'informazione e l'educazione permanente. Tutto ciò richiede investimenti e finanziamenti: non è credibile, non è possibile sostenere tutto ciò «senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica». Ci sono proposte in campo, emendamenti proposti anche dal Partito Democratico, che indicano una strada: vedremo dunque l'atteggiamento della maggioranza alla prova dei fatti. Tuttavia, occorre saper guardare avanti: l'equilibrio dei sistemi pensionistici è una cosa seria ed il loro rapporto con gli andamenti demografici richiede soluzioni complesse da mettere in campo nel breve e nel medio periodo. È per questo che è difficile parlare, ad esempio, di donne e pensioni, di donne e lavoro, senza nel contempo saper creare le condizioni per una sostenibilità sociale vera dei cambiamenti che si vogliono realizzare e per una vera parità. forse si risolvono alcuni problemi finanziari, ma si rischia dì strappare le relazioni sociali del Paese, e non so quale sia il male peggiore. Occorre, mentre si interviene, sostenere la famiglia e la natività, ma occorre soprattutto creare nuovi posti di lavoro realmente accessibili anche alle donne: unica vera soluzione per sostenere i futuri equilibri dei pur diversificati sistemi pensionistici. Occorre sostenere l'integrazione regolare di nuovi cittadini che possono concorrere al riequilibrio demografico e spesso coprono segmenti lavorativi scarsamente appetibili. Per affrontare seriamente e con civiltà tali problemi, che hanno carattere epocale, bisogna sempre aver presente che stiamo ragionando non di numeri e di statistiche, ma di donne e di uomini, con pari dignità e diritti. Sono presenti in tribuna e assistono ai lavori durante la loro visita al Senato gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Riccati-Luzzatti» di Treviso. A loro e ai loro insegnanti va il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio.

offre a tutti noi spunti di riflessione su materie ampie e su vaste scelte che, in prospettiva, dovremo fare e che il Governo dovrà poi realizzare.

La parità la vediamo scritta in tante carte, in tanti documenti e in tante norme, ma non riusciamo poi a vederla realizzata, se non in minima parte. Quest'ultima direttiva sulla parità a me pareva fosse

legata al benessere, grazie a un sistema di servizi sociosanitari che ha consentito al nostro Paese di guadagnare attese di vita da record mondiale.

di recupero sociale e soprattutto economico, rivestono un ruolo fondamentale. Pertanto, potremmo

per rimodellare l'asse dello scambio lungo cui sono disegnate le traiettorie pensionistiche, bilanciando l'impatto del ritardato abbandono del servizio non con il freno della progressività, ma con l'acceleratore dei servizi compensativi all'onerosità sociale implicita nella condizione della donna lavoratrice. si potrebbe aprire un confronto con le organizzazioni sindacali, per definire un cantiere di sperimentazione socio-contrattuale, dove le donne ritardino il tempo del pensionamento in relazione all'intensità delle misure di agevolazione nell'organizzazione della loro vita personale e familiare. spiegare ancora meglio il concetto che sta alla base e la filosofia che ispira alcuni emendamenti presentati in questo senso dalla maggioranza e dall'opposizione.

è e sarà sempre più importante e determinante per motivi demografici, economici e - consentitemi di dirlo per il mio modesto punto di vista - per quella partecipazione da protagoniste che dobbiamo poter avere sempre: quando siamo giovani ed entriamo nel mercato del lavoro, quando fatichiamo tanto a restarci e quando alla fine ne usciamo e rischiamo di farlo con la scusa di un risarcimento, in realtà più più povere e meno forti, e quindi più vulnerabili, proprio nella fase più delicata della nostra vita. Allora cosa emerge? Che se c'è una modulazione vera da fare non è la progressione automatica, non è il bieco calcolo di contributi e di pensionamento. Voglio ricordare che noi da oltre dieci anni viviamo all'interno di un modello pensionistico previdenziale contributivo e non più retributivo e ciò determina che le pensioni che noi percepiremo - mi riferisco alle donne della mia generazione, per esempio - saranno calcolate solo ed esclusivamente sulla base dei contributi realmente versati e, mi consenta, Presidente, cinque anni di contributi in meno pesano, e come, su una pensione. Allora, dicevo, dove va fatta la rimodulazione con serenità, con onestà, con la giusta rappresentanza degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori? Guardando al loro vero interesse e non a bandiere ideologiche, va fatta misurando e mettendo a confronto, là dove ci sono (quali, quanti e come sono fatti), quei servizi sociali che lo Stato e gli enti locali devono garantire alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Là dentro possiamo trovare probabilmente la soluzione per ricomprendere da protagoniste le donne all'interno del sistema produttivo, sia pubblico sia privato. In questo caso specifico, poiché ci limitiamo a parlare del settore pubblico, sono certa che da quelle donne che lavorano per lo Stato, per gli enti locali e per tutto il sistema della funzione pubblica, e lo fanno, all'interno della crisi che viviamo, in una condizione di serenità, di contrattualità

proprio da quelle donne protagoniste del processo di modernizzazione della nostra amministrazione pubblica e della nostra burocrazia possiamo ricevere un ulteriore insegnamento e un ulteriore contributo alla crescita economica di questo Paese. Una crescita che non passa dalla loro pensione: passa dalla loro partecipazione attiva a quella società la cui pubblica attiva a quella società la cui pubblica amministrazione è leva di sviluppo e di competitività e non una palla al piede da trascinare. Se quindi, all'interno del recepimento della direttiva sulla parità, noi possiamo fare alcune riflessioni importanti, una di queste riguarda il trattamento pensionistico e molte altre riguardano l'occupazione delle donne, il sostegno all'ingresso nel mercato del lavoro, quel sostegno a poter restare dentro questo mercato e a conciliare la loro vita lavorativa con quel

non c'è soluzione nazionale alla crisi. Anzi, qualunque tentativo di soluzione nazionale risulta semplicemente controproducente, magari buona per i titoli dei giornali ma certamente controproducente a medio termine.

del Partito Democratico, avere sollevato questo problema da molti mesi a questa parte. I colleghi senatori e le colleghe senatrici troveranno questa mattina in casella un simpatico libretto, frutto del convegno al quale molte di voi hanno partecipato, ho voluto dare un titolo non scherzoso, ma certamente diretto. Si intitola "Pensionata sarà lei", ed è accompagnato da una lettera. L'ho voluto fare non perché gli interventi a quel convegno fossero tutti favorevoli. Al contrario! Ci sono stati interventi da parte sindacale e non solo di grandissima resistenza per quanto riguarda l'equiparazione dell'età pensionabile che, peraltro, è un atto dovuto: dovremo farlo. La cosa fantastica è che - mi sembra di capire - persino la proposta della collega Bonfrisco di una delega al Governo di 18 mesi non sarà accettata, a

Il problema è politico, non procedurale. La Commissione bilancio, per esempio, dà parere contrario a tutta una serie di emendamenti, che mi parevano invece di indirizzo molto importante sul recepimento della direttiva n. 54, perché "costano".

di consultare? Avevamo l'opportunità straordinaria di affrontare la questione dell'accesso al mercato del lavoro femminile nel nostro Paese su un binario equilibrato,

attenzione ai tempi flessibili, persino alla maternità; dall'altra, contestualmente, risolvendo un problema che ci fa notare l'Europa sull'innalzamento dell'età pensionabile, essendo inteso peraltro che, come avvenuto in altri Paesi, quei risparmi dovevano essere dedicati - questo dicevano gli emendamenti - a quel fondo di conciliazione - chiamatelo come volete - per cominciare a risolvere una questione patetica in Italia La questione è che le donne ed il mondo femminile in Italia sono il surrogato di tutti quei servizi sociali che non ci sono,

Siamo delle funambole e, ovviamente, questa situazione a molta parte del corpo politico sociale italiano fa grandemente comodo.

i figli di mio figlio, che ha adesso 60 anni, li alleva una badante rumena. Però siamo sempre lì, va a finire che in Italia le donne un lavoro non lo cercano neanche. Se al Nord

Questa è la società italiana, non è solo la politica. Quante sono le rettrici di università in Italia? Due. Quante sono le direttrici di banca? Zero. Quante le direttrici di giornali quotidiani? Due. E avanti di questo passo. Ma procedendo di questo passo, onorevoli colleghi, c'è una responsabilità in più della politica, che non può essere quella lamentosa e di pura constatazione di una fotografia impietosa (quella l'avevamo già fatta con la Nota aggiuntiva di Lisbona che nessuno dei Governi ha mai brillato molto sul punto, però i tempi cambiamo e credo che, nella situazione in cui ci troviamo, penalizzare il patrimonio femminile sia una responsabilità grave. grave. Questa era un'occasione che potevamo cogliere insieme, peraltro, ma mi sembra di avere capito che non è più tempo neanche questa volta. Non so quando sarà mai il tempo. Onorevoli colleghe, sono convinta che nessuno ci farà spazio se non ce lo prendiamo, né qui, né nella società.

di tanta attività e di tanta presenza di colleghe senatrici non manderebbe sicuramente un buono messaggio alle donne italiane. Capisco, ci sono le elezioni, ma insomma, in una democrazia si vota ogni anno, se guardiamo alle elezioni non andiamo da nessuna parte. Mi auguro quindi che gli interventi svolti si traducano in posizioni coerenti quando arriveremo alla votazione degli emendamenti.

Signor Presidente, con il disegno di legge n. 1078 il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione della legge comunitaria, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta legge Buttiglione), che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, individuando nella legge comunitaria lo strumento normativo cardine diretto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario. Strumento normativo cardine, anche se non esclusivo: infatti, il provvedimento che oggi esaminiamo riproduce in gran parte il contenuto dispositivo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 approvato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio 2008, presentato in Parlamento il successivo 26 febbraio, che ha visto interrompersi il proprio *iter* di approvazione a causa dello scioglimento delle Camere. Dal testo sono state stralciate le disposizioni che, nelle more della ripresa dell'ordinaria attività parlamentare, hanno trovato collocazione in altri testi normativi. Nello stesso tempo si è provveduto ad aggiornare il contenuto del disegno di legge, sia attraverso l'integrazione degli allegati contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, sia attraverso l'inserimento di nuove disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale

direttive attuate e da attuare per via amministrativa e quelle da attuare per via regolamentare, giustificando le ragioni dell'avvenuto mancato inserimento di direttive i cui termini di recepimento sono scaduti o in scadenza, fornendo l'elenco degli atti normativi con i quali le singole Regioni e Province autonome hanno dato attuazione alle direttive nella materie di loro competenza. Il disegno di legge comunitaria 2008 mantiene in gran parte la struttura delle precedenti leggi comunitarie e, al tempo stesso, conferma le importanti novità previste dalla legge comunitaria

anche su altri punti, però non posso esimermi dall'affrontare la questione delle pari opportunità. L'articolo 11 (8 nel testo del Governo) modifica il termine della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che riguarda l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, per adeguarlo al termine di riferimento che l'articolo 30-*ter* della direttiva prevede nel caso di difficoltà di attuazione. Il Governo è delegato ad attuare, entro il 15 agosto 2009, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva

La direttiva cosiddetta di rifusione concerne la parità di trattamento in materia di remunerazione, di regimi professionali e di sicurezza sociale, di accesso al lavoro, alla promozione ed alla formazione professionale, e di condizioni di lavoro. contenute riguardano in primo luogo l'adozione da parte degli Stati membri di misure che garantiscano la tutela giurisdizionale e il diritto di parità e di trattamento, nonché forme di risarcimento e di riparazione del danno. In tale ambito, va ripreso il principio dell'onere della prova in base al quale la parte convenuta dovrà provare l'insussistenza della violazione, laddove la parte lesa avrà prodotto elementi sufficienti a far ritenere che si sia verificata una forma di Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento, gli Stati membri dovranno quindi designare uno più organismi incaricati, tra l'altro, di prestare assistenza alle vittime delle violazioni, per svolgere opportune richieste ed adottare misure in favore del dialogo tra le parti sociali e con le organizzazioni non governative e stabilire norme atte a proteggere i lavoratori da trattamenti sfavorevoli che costituiscono una reazione ad una richiesta di rispetto del principio di parità di trattamento. Dico questo, e sarebbe lunga l'elencazione, perché non volevo soltanto riaffermare quello che hanno sostenuto le colleghe che mi hanno

annuale delle Nazioni Unite di New York, alla quale ho avuto l'onore di partecipare in rappresentanza del Senato. Ebbene, i temi trattati

la questione dell'occupazione. Allora, è evidente che mentre discutiamo della legge comunitaria e nel momento in cui recepiamo questa importante direttiva europea europea non ci possiamo esimere dal trattare tali argomenti. Inoltre, non possiamo non tener conto della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alla pensione di vecchiaia.

finalizzate al riordino della normativa in materia di sistema pensionistico e volte a consentire la cooperazione su un base volontaria dell'età pensionabile tra uomini e donne. Tale ordine del giorno, giorno, contestualmente, chiede al Governo che le maggiori entrate derivanti da tali misure vengano utilizzate per la creazione di una rete integrata di servizi necessaria per sostenere le esigenze delle madri lavoratrici e favorire iniziative legislative

parlare di condivisione di responsabilità tra uomini e donne e non solo di pari opportunità è il vero cambiamento, perché quella delle pari opportunità è una questione ben conosciuta dalla pubblica opinione e ormai radicata nella struttura sociale dei Paesi democratici.

ricordare che la disciplina, palesemente modellata sulle società di capitali quotate, è totalmente incompatibile con le attuali caratteristiche delle società cooperative. Dunque, è molto importante il recepimento da parte del Governo dell'emendamento con il quale si è introdotto, all'articolo 30, uno specifico criterio di delega relativo all'attuazione della suddetta direttiva, con il quale si prevede espressamente che le disposizioni non si applicano alle società cooperative. Si salvaguarda in tal modo il modello funzionale organizzativo delle società cooperative esercenti attività bancaria, come le banche di credito cooperativo e quelle popolari, preservandone i caratteri strutturali come il voto capitario, eliminando il numero delle deleghe che possono essere rilasciate, e l'operatività a sostegno dello sviluppo delle autonomie locali, tanto più necessaria alla luce dell'attuale scenario macroeconomico. In conclusione, il provvedimento è di grande rilievo per la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione comunitaria. È quindi importante che quest'Aula si renda conto che la materia comunitaria costituisce ormai un pilastro

se la 14a Commissione del Senato, così com'è, sia utile in riferimento alle questioni che solleviamo con la legge comunitaria e a quali condizioni;

In ultimo, rispetto al tema dei servizi (mi rivolgo anche ai colleghi che si occupano di amministrazione locale),

sul fatto che i partiti europei debbano essere trasparenti e proporre una Presidenza che duri due anni e mezzo; sul fatto che la Presidenza Obama ha cambiato le condizioni, indipendentemente dai colori politici, perché chiede all'Europa una

quando arriveremo al momento delle elezioni europee e, possibilmente, avendo già in previsione il cambiamento e la possibilità di discutere di quello che accadrà il prossimo anno, alla fine di quello in corso, a novembre. Allora la legge comunitaria - e concludo veramente, signor Presidente - sarà divenuta un atto non di mera riproposizione

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, i temi trattati nel disegno di legge n. 1078 sono tanti e tutti meritevoli di una maggiore attenzione da parte di quest'Assemblea. Essi riguardano diversi settori del nostro vivere quotidiano ed incidono significativamente sul tessuto sociale del Paese. Cito, ad esempio, i temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'esercizio delle attività televisive e della parità di genere in materia di lavoro. riguardo, si sono dilungate altre colleghe e, quindi, io rinuncio a farlo, rilevando però che non si può costruire la parità partendo dalle pensioni. Sono necessari interventi anteposti a questo. Il concetto di carattere generale che vorrei sottolineare è la necessità che ci sia una maggiore consapevolezza nella gente, ma soprattutto nella classe politica, rispetto alla nostra appartenenza europea, con tutto ciò che ne consegue. Il recepimento delle direttive europee e l'adempimento degli obblighi comunitari non sono - come già ha detto la senatrice Bonino - degli *optional*, che si prendono se fanno comodo; non sono nemmeno contentini che si danno a qualche burocrate a Bruxelles, come qualcuno ha scritto. Rappresentano, invece, uno degli elementi del nostro stare insieme in Europa della politica comune europea, che va rafforzata e valorizzata, tanto più nei momenti di crisi, come quella attuale, ma anche in vista dell'allargamento dell'Unione verso nuovi Stati. Mi piacerebbe che l'azione politica italiana fosse maggiormente contaminata dall'ottica europea, ma forse - me lo auguro - avremo modo di confrontarci su questi temi nell'imminente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Con il mio intervento desidero porre l'attenzione su una problematica specifica, inserita nel Capo III del disegno di legge, e cioè l'attuazione del regolamento relativo al cosiddetto GECT (gruppo europeo di cooperazione territoriale). Me ne sono occupata fin dall'approvazione del regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel 2006. Provenendo da una Regione di confine, non posso che esprimere soddisfazione, perché anche nel nostro Paese si concretizza finalmente la possibilità di costituire i GECT, uno strumento di cooperazione a livello comunitario, che aiuterà gli Stati membri nel campo della cooperazione transfrontaliera. L'obiettivo del GECT è quello di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale e rafforzare così la coesione economica e sociale. Vorrei ricordare, a questo proposito, che la Slovenia ha già approvato il regolamento, che per il Friuli-Venezia Giulia può rappresentare inoltre un supporto nel processo per la creazione dell'euroregione - di cui si parla da anni, ma che negli ultimi tempi un po' sbiadita - intesa come forma di cooperazione stabile e rafforzata tra territori appartenenti a Stati nazionali diversi. Nonostante quest'attesa, nella Regione Friuli-Venezia Giulia la cooperazione transfrontaliera è una realtà assodata. In questi anni, attraverso i fondi Interreg ed altri fondi europei, sono stati realizzati moltissimi progetti che hanno coinvolto le imprese, i servizi, la salvaguardia del territorio, le infrastrutture, la cultura ed altro. Per una Regione circondata da confini, che fortunatamente di recente sono stati abbattuti, la cooperazione transfrontaliera è come il pane quotidiano: non se ne può fare a meno, attraverso di essa si può progettare un futuro di sviluppo economico e sociale, ma soprattutto di pace. Attraverso la cooperazione territoriale che il GECT favorirà, in quanto dotato della più ampia capacità giuridica, si riesce a rinsaldare amicizie, a rafforzare la convivenza tra identità, lingue e culture diverse e a guardare con fiducia il proprio futuro nella casa comune europea. I GECT - e mi auguro che non sopravvengano difficoltà o ostacoli vari per la loro autorizzazione - offrono l'opportunità di partire dal basso, dalle piccole cose e da piccoli progetti, che coinvolgano soggetti pubblici altrimenti in difficoltà ad utilizzare i fondi europei. Si dovrà fare attenzione perché non si sovrappongano ad altri enti e non diventino l'ennesimo organismo pletorico. A me sembra che, proprio sul confine orientale, la creazione dei GECT transnazionali possa contribuire anche a rimuovere i rancori del passato, che purtroppo ogni tanto riemergono dolorosamente, come abbiamo potuto constatare recentemente. Alcune positive esperienze di GECT ci sono già nei diversi Stati membri: anche nel Friuli-Venezia Giulia vi sono alcune idee e progetti: spero che, con l'approvazione di questo disegno di legge, possano realizzarsi in tempi brevi e, nello stesso tempo, mi auguro che possano rappresentare il passo decisivo per la costituzione della nostra Euroregione.

di un lavoro importante, perché senza questi interventi il nostro Paese andrebbe incontro a sanzioni, sia di da parte dell'Unione europea. Le prime consisterebbero in una serie di procedure che indicherebbero che il nostro Paese non ha adempiuto a questa

però questo provvedimento mi viene in mente un'ulteriore riflessione. Solo quest'anno - perché abbiamo una legge comunitaria tutti gli anni e molte norme europee vengono recepite in altri provvedimenti, non necessariamente nella legge comunitaria, che ne accoglie soltanto la maggior parte - vi sono ben 125 pagine di testo. pagine di testo. Molti degli articoli sono rappresentati da deleghe che, dunque, daranno vita a decreti legislativi, a decreti ministeriali, a regolamenti e a tutta una serie di norme,

veramente indispensabile che l'Unione europea inondi gli Stati membri, i Governi e - ciò che più conta - le imprese e i cittadini, con tutte queste norme.

E forse non è del tutto casuale il fatto che l'Unione europea accusi da molto tempo una crescita inferiore a quella di altri Paesi, che trovandosi liberi dalle norme imposte

È vero che è difficile aspettarsi questo da istituzioni europee un po' complicate. Noi, ad esempio, stiamo discutendo di differenziare i ruoli delle nostre due Camere, che spesso compiono lo stesso lavoro, ma le istituzioni europee riescono nel capolavoro di avere una sola Camera, una sola Camera, con due sedi, perché bisogna ricordare le ambizioni della piccola città di Strasburgo, che vuol essere al contempo capitale europea, ma poi non lascia costruire un aeroporto di degne dimensioni per cui risulta difficilissima da raggiungere.

voglio innanzitutto esprimere soddisfazione per essere finalmente arrivati alla discussione in Assemblea della legge comunitaria per il 2008. Questa legge comunitaria è frutto di un lavoro condiviso tra maggioranza ed opposizione, come ho potuto constatare dal momento che il testo che abbiamo analizzato è stato inizialmente redatto dal Governo precedente e poi ripresentato all'esame parlamentare in Commissione. Come Italia dei Valori, abbiamo accolto con favore alcune proposte del relatore e del Governo e, allo stesso modo, alcuni nostri emendamenti sono stati recepiti, mentre altri sono stati ripresentati in Aula, nella speranza che, considerato

ricorda come il nostro ordinamento sia gerarchicamente vincolato alle disposizioni comunitarie, in virtù dell'articolo 11 della nostra Costituzione e di tanta recente giurisprudenza, la quale ha sancito il primato delle norme europee su quelle ordinarie nazionali. Lo strumento della legge comunitaria dovrebbe pertanto rappresentare, per il nostro Paese, una sorta di finanziaria europea, ossia lo strumento principale con cui programmare un anno di interventi normativi.

sia delle raccomandazioni della Commissione che degli indirizzi del Consiglio e del Parlamento europeo, tramite la trasformazione di questi in politiche nazionali concrete. comunitaria apparterrebbe all'area delle leggi a contenuto vincolato, una delle materie che non può essere oggetto di *referendum* *ex* articolo 75 del testo costituzionale, come le leggi di bilancio o le ratifiche di trattati internazionali. ancora, nella nostra cultura politica, essa non riceve l'attenzione che merita, in quanto la sua discussione è spesso compressa da altre esigenze interne e l'oggetto proprio della legge viene sovente usato strumentalmente come contenitore per procedere a riforme che sono interesse della maggioranza del momento. In merito ai tempi parlamentari, vorrei ricordare che il processo di approvazione del provvedimento in esame è stato davvero lungo, considerando che il Ministro per le politiche europee, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie e della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sarebbe tenuto a predisporre il disegno di legge e a presentarlo al Parlamento

Per questo auspico che nel futuro si possa procedere con maggiore celerità e nel rispetto dei tempi fissati dalla legge La Pergola e poi dalla legge Buttiglione. L'Italia dei Valori è un partito profondamente europeista, che vede nella Comunità una risorsa e un'opportunità preziosissima per lo sviluppo del nostro Paese, e che tiene a garantire il nostro impegno nel progetto federale del quale facciamo parte sin dal Trattato di Roma del 1957 e sin dalle proposte costruttive di Altiero Spinelli. Pertanto, verso la legge comunitaria abbiamo mostrato un atteggiamento pienamente collaborativo. Tuttavia, non potevo esimermi dal fare queste considerazioni sui tempi di approvazione, come non posso non portare alla vostra attenzione, cari colleghi, che anche in merito al contenuto della legge diversi aspetti appaiono a noi molto critici: sia perché diverse disposizioni introdotte in via emendativa risultano estranee alla materia della legge, sia perché in altri punti, anche su materie sensibili, si è delegato il Governo a legiferare con eccessiva genericità, sia, infine, per l'atteggiamento discrezionale con cui la maggioranza ha deciso quali sentenze dell'Unione europea recepire e quali no. Si sa, la legge comunitaria è comunque fatta da un Governo nazionale, e viene discussa e approvata da un Parlamento nazionale, pertanto siamo consci che di riflessi nazionali si vestano i criteri con cui si selezionano le priorità, e a tal tal proposito mi rivolgo al Governo con uno spirito di criticità. Esempio di tale influenza è stata la scelta di recepire la decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze penali fra Stati membri dell'Unione europea, contenuta nell'articolo 49 del disegno di legge n. 1078. legge n. 1078. Nella relazione illustrativa all'emendamento che accelera di un anno l'attuazione inizialmente prevista per il 2011, il Governo spiega come l'urgenza di recepire sia stata posta dai recenti fatti di cronaca e dai dati emergenti circa il numero di cittadini comunitari detenuti nelle carceri italiane, che ammontano ad oggi a 4.000 unità. Come Italia dei Valori abbiamo riconosciuto il merito di tale decisione quadro e la correttezza la correttezza di procedere ad una rapida attuazione, poiché lo strumento, da un lato, permette di diminuire il numero di detenuti per il nostro sistema carcerario, e, dall'altro, permette ai condannati di scontare la pena detentiva in condizioni più favorevoli, ossia

una delucidazione sullo stato di attuazione dello strumento. Infatti, caro Ministro, se la legge quadro non viene ugualmente recepita dagli altri Stati membri, perde ogni operatività, poiché l'efficacia si basa sulla cooperazione fra autorità giudiziarie, e rimane soltanto un atto normativo vuoto con una valenza più demagogica e politica

dell'*iter* di recepimento della Romania, poiché proprio a tale Paese ci si riferisce quando il Governo parla di attualità e dati, se si considera che il 73 per cento dei detenuti comunitari nelle carceri italiane è romeno, come si evince dalla relazione del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Se davvero lo strumento divenisse operativo entro un anno, l'Italia dei Valori non potrebbe che considerarlo positivamente, poiché la decisione è in linea con la politica che da sempre perseguiamo, ossia il contemperamento fra libertà e solidarietà. Tuttavia, non si può dire lo stesso per altre disposizioni contenute nell'articolato del disegno di legge n. 1078. Appare controversa, ad esempio, l'operazione fatta dal Governo all'articolo 24, ove, con un emendamento di ben 29 pagine, che titola "Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie", si va a modificare estensivamente l'intera disciplina tributaria e, sotto il profilo contenutistico, si regolano aspetti assai distanti fra loro come, ad esempio, il regime sui dividendi, la revisione in materia di tabacchi o, ancora, la disciplina dei giochi pubblici. Oltretutto a tale norma si trova la copertura economica necessaria sulla base di previsioni assolutamente aleatorie circa l'emersione del gioco illegale, procedendo pertanto ad una delle solite norme che stabiliscono il "cosa", ma non definiscono il "come". "come". Altro punto che deve necessariamente essere messo in luce come errato utilizzo dello strumento comunitario è l'aver inserito nell'allegato B, fra le direttive da recepire, la n. 115 del 2008, ossia la cosiddetta direttiva rimpatri, senza che venga esplicitato nessun tipo di criterio o principio di delega. Cari colleghi, la semplice inclusione in allegato di una norma comunitaria da recepire può avvenire solo qualora la sua applicabilità sia praticamente diretta, non necessiti di modifiche al nostro ordinamento interno e non presupponga una interpretazione del testo. La direttiva rimpatri non fa certo parte di questa categoria di norme, anzi, è una disposizione controversa, assai osteggiata dal PSE, dai Verdi e dall'ALDE in fase di dibattito al Parlamento europeo, ed è stata formulata come una sorta di pacchetto di compromesso che lascia amplissima discrezionalità agli Stati membri per scegliere come e cosa applicare di quanto dispone in materia di ritorno volontario degli immigrati illegali, durata e condizioni di detenzione temporanea, trattamento dei minori non accompagnati, divieto di reingresso. Ad esempio, fissa la permanenza degli immigrati nei CPT (centri di permanenza temporanea) per un massimo di sei mesi, ma lascia liberi gli Stati membri di prolungarlo di altri dodici. Il Governo cosa ha fatto? Da una parte ha anticipato alcune disposizioni come quella sui CPT nel decreto Maroni, dall'altra ha drasticamente inserito la direttiva nell'allegato B e lo ha fatto tramite un emendamento sul quale io ed i colleghi non abbiamo avuto modo di discutere,

che da una parte si è tenuto il rigore e si sono accelerati i tempi, ma dall'altra si è optato per l'estrema discrezionalità nel selezionare quali sentenze della Corte di giustizia recepire (parleremo anche di Europa 7).

Colleghi, vorrei farvi presente che è stata disattesa la pronuncia della Corte di giustizia con la quale la giurisprudenza europea ha sancito l'illegalità della penalizzazione fatta a Europa 7 per privilegiare Rete 4 nella distribuzione delle frequenze televisive. pertanto che, ora che andremo ad analizzare i nostri emendamenti e i nostri ordini del giorno, questi vengano interpretati nel giusto spirito costruttivo con il quale sono formulati, ossia per armonizzare virtuosamente le leggi italiane con quelle europee, anche laddove queste vadano ad inficiare gli interessi del Governo. Vorrei concludere condividendo quanto ha detto la presidente Bonino; il discorso in 14a Commissione riferito alla direttiva 2006/54/CE e alla sentenza della Corte di giustizia

corso del mio intervento mi soffermerò soltanto sulla relazione relativa all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Altri colleghi hanno avuto modo di intervenire sulla Legge comunitaria e di

A questo proposito voglio sottolineare l'eccellente lavoro fatto dalla ex ministro Bonino, che ha permesso al nostro Paese - non ad una parte politica - di recuperare credibilità nei confronti delle istituzioni europee con riferimento all'intera partita delle infrazioni e anche in materia di ottemperanza rispetto all'ordinamento europeo. Credo che sia un risultato importante per l'immagine del Paese Paese e per le istituzioni italiane, che non va sprecato o comunque non va fatto oggetto delle contrapposizioni tra maggioranza e opposizione.

con un processo complesso che poi si cala, attraverso gli strumenti legislativi europei, nel diritto nazionale. Se il procedimento è abbastanza macchinoso, lungo e complesso,

due momenti importanti, essenziali nella vita del Parlamento, di discussione e confronto sulla politica e sulla legislazione europea, scindendo la Relazione annuale sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea dalla legge comunitaria. Sono due momenti importanti che tendono a responsabilizzare sempre di più le Assemblee nazionali e soprattutto

Queste sono in sostanza le questioni e i propositi che mettiamo in rilievo nella proposta di risoluzione

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, vorrei fare innanzitutto una osservazione al riguardo dell'articolo 41 della legge comunitaria 2008 alla nostra considerazione, che conferisce al Governo delega per l'attuazione dell'importantissima direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. Mi chiedo se i criteri e princìpi direttivi indicati tutelino a sufficienza il cittadino italiano. Per essere più chiaro, mi riferirò al caso dei servizi di ingegneria, che conosco. Coloro che nel nostro Paese fruiscono di questi servizi, quali la progettazione strutturale di un ponte o di un edificio, la direzione dei lavori o il collaudo di opere civili, servizi, per inciso, di elevata qualità intellettuale, servizi per cui la legge prescrive la firma di un ingegnere iscritto ad albo professionale con adeguate qualifiche (tra cui il superamento dell'esame di Stato), sono stati finora ben tutelati nel nostro Paese, sia sotto il profilo della qualità della prestazione professionale, sia sotto il profilo delle norme deontologiche a cui l'ingegnere deve conformare il suo comportamento. In particolare, mi sembra che il testo del principio e criterio direttivo *f)* dell'articolo 41, che consente allo Stato di imporre requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi in presenza di giustificati motivi, signor tra questi l'esigenza della sicurezza delle strutture e dei manufatti, che pure costituisce un interesse primario della società. Inoltre, non mi pare sufficientemente preciso il criterio direttivo Il principio di garantire una effettiva parità ai cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea è sacrosanto. Ma come ottenere questa parità? Il criterio direttivo *s)* al riguardo non precisa nulla. A mio avviso sarebbe invece stato opportuno richiamarsi all'interesse primario dei cittadini, fruitori dei servizi. In base a tale interesse primario la prescritta equiparazione in molti casi dovrebbe essere attuata non rendendo meno restrittiva la disciplina per i cittadini italiani prestatori di servizio, ma vincolando a più severi requisiti i cittadini di altri Paesi dell'Unione europea che intendono svolgere servizi in Italia. Per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007, un testo di 395 pagine, presentato al Parlamento dal ministro per le politiche europee Emma Bonino il 31 gennaio 2008, mi limiterò a due osservazioni. La prima osservazione riguarda le gravi carenze della Relazione. Prima di tutto, in essa risulta assai difficile orientarsi, data l'assenza di adeguati inquadramenti storici, che forniscano sui vari argomenti almeno alcuni cenni su quanto fatto o impostato negli anni precedenti. Altro cospicuo suo difetto è di essere praticamente priva di considerazioni critiche. I fatti, le azioni, le iniziative, eccetera, vengono presentate senza che su di esse vengano espresse valutazioni e giudizi. Ciò è veramente singolare in una sede di valutazione politica come quella della Relazione. Il sentimento prevalente nella Relazione è quello di un apprezzamento tacito e generale di tutte le azioni intraprese dalla Commissione e dall'Unione europea, un sentimento sostanzialmente enfatico. Domande del tipo: «Conviene all'Italia?», oppure: «L'Italia risulta svantaggiata?», non vengono mai poste su nessuna iniziativa. La Relazione presenta inoltre vistose mancanze. Ad esempio, nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Relazione non informa sull'avanzamento del VII Programma quadro di ricerca in particolare sulla partecipazione italiana a tale programma), non dice nulla sul programma di ricerca nel settore della fusione nucleare, non menziona le azioni fatte in campo spaziale. Sorprende la mancanza di raccordo tra questa Relazione e le precedenti. Ad esempio, la Relazione non menziona in nessun modo né il programma di cooperazione culturale pluriennale denominato «Cultura 2007» (citato come importante nella Relazione per l'anno 2004), né il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, denominato PICO, per cui addirittura, nella Relazione per l'anno 2005, si diceva che i Governi sono tenuti a fornire rapporti annuali sullo stato di attuazione. La ragione di questi disequilibri della Relazione, di queste omissioni, della mancanza di valutazioni critiche, eccetera è dovuta alla sua frettolosa modalità di redazione, risultante dalla giustapposizione *tout court* delle relazioni dei Ministeri, a loro volta assemblate semplicemente come collazione degli *output* dei direttori generali, i quali certamente non si dilungano su quello che la loro direzione non ha fatto (e avrebbe dovuto fare) e non si preoccupano affatto di inquadrare le loro azioni dal punto di vista storico; men che meno si azzardano ad esprimere valutazioni critiche. Speriamo che la Relazione dell'anno prossimo non presenti più tali anomalie. seconda osservazione riguarda la politica dell'energia. Per questa politica l'anno 2007 è certamente stato di estrema rilevanza. Il Consiglio europeo di primavera, l'8-9 marzo 2007, ha infatti approvato all'unanimità il noto pacchetto «energia-ambiente 20-20-20», proposto dalla Commissione europea. Al contrario di quanto si legge nella Relazione, a pagina 277, il suddetto pacchetto «20-20-20» non deriva affatto dal Libro verde «Una strategia europea per una energia sostenibile competitiva e sicura», presentato nel marzo 2006. Questo Libro verde, infatti, non prevedeva nessun obiettivo vincolante, si ispirava alla consueta filosofia europea di un equilibrato gradualismo e postulava interventi per far fronte ai cambiamenti climatici solo in termini generici. Nel gennaio 2007 compare invece un documento della Commissione che contiene una proposta che non è esagerato definire rivoluzionaria, con la configurazione dei noti, estremamente ambiziosi, obiettivi vincolanti, da conseguire entro il 2020. A proposito di questa radicalizzazione della politica energetica europea, dispiace che tra il momento del suo annuncio, come proposta della Commissione europea, effettuato nel gennaio 2007, e la sua deliberazione nel Consiglio europeo di primavera, siano intercorsi a stento quaranta giorni. Non c'è stato quindi tempo per i Parlamenti nazionali di esprimere al riguardo una qualche opinione. Una tale modalità di formulazione di obiettivi vincolanti per l'Unione europea è lesiva di fondamentali diritti dei cittadini e dei Parlamenti nazionali; per decisioni così rilevanti non è ammissibile la politica del blitz. Questa radicale e costosa innovazione della politica energetica comunitaria è stata presentata come urgentemente necessaria per rallentare il riscaldamento globale in atto, attribuito in gran parte all'anidride carbonica prodotta nei processi di combustione dei combustibili fossili. Ma tale attribuzione non è condivisa da una parte consistente di climatologi, che ritengono importanti anche altre cause, tra cui cause naturali, come le variazioni dell'attività del sole e l'influenza di attività umane, quali l'agricoltura, l'estesa urbanizzazione, la deforestazione e l'inquinamento dell'atmosfera con fumi ed incendi. L'anidride carbonica non è un gas inquinante dell'atmosfera: è per suo merito che esiste la vita sulla terra. L'effetto serra prodotto dall'anidride carbonica è pari solo ad un terzo di quello, nettamente prevalente, del vapore acqueo e delle nuvole, ed è già abbastanza in saturazione, come effetto serra, alle concentrazioni Tra i tre obiettivi vincolanti, quello nettamente più gravoso riguarda il conseguimento entro il 2020 di una quota di consumi energetici finali da fonti rinnovabili non inferiore al 20 cento dei consumi energetici finali complessivi. Per l'Italia, come sappiamo, tale obiettivo è stato poi ridotto al 17 per cento nel *burden sharing agreement* dello scorso dicembre. Si tratta sempre, tuttavia, di un obiettivo pressoché irraggiungibile. La poderosa incentivazione pubblica di alcuni comparti industriali interessati alla produzione delle energie da fonti rinnovabili determinerà lo sviluppo in Italia di un settore industriale di una certa importanza, la cui vita non dipende da una reale richiesta di mercato, ma dalla sua incentivazione. La decisione dell'Unione europea sta cosi determinando lo sviluppo di un settore industriale assistito, che ovviamente peserà in futuro sui decisori pubblici per continuare a godere di condizioni di favore. Questa forte incentivazione delle energie rinnovabili, il cui onere è valutato per l'Italia in svariati miliardi di euro all'anno per il periodo 2013-2020, sarà a carico della bolletta elettrica. Il prezzo del chilowattora è quindi destinato ad aumentare in futuro, e non poco. Tale aumento sarà diverso per ogni Paese dell'Unione europea, a seconda della particolare incentivazione a carico della bolletta elettrica che verrà decisa in quel Paese. La disposizione in questione determinerà, quindi, una rilevante distorsione delle economie dei vari Paesi e della relativa competitività. L'aumento del prezzo del chilowattora sarà particolarmente elevato nel nostro Paese per le intrinseche maggiori difficoltà a ricorrere alle energie rinnovabili che esso ha rispetto agli altri Paesi europei. Si determinerà così in Italia una minore competitività del sistema produttivo e quindi la perdita di posti di lavoro. La decisione del pacchetto clima-energia assunta dal Consiglio europeo di primavera, nel marzo 2007, causerà quindi per il nostro Paese varie conseguenze negative, quali un considerevole aumento del prezzo del chilowattora, la creazione di un settore industriale assistito, una rilevante perdita di competitività, anche nei riguardi degli altri Paesi europei, la perdita dì posti di lavoro. Il tutto senza che vi sia sufficiente motivazione per assoggettarci a simili privazioni.